dopo il lungo e articolato dibattito di ieri mi preme prima di tutto precisare che la bozza di questo disegno di legge è stata predisposta dal Comitato 3 ottobre, presieduto da Tarek Brhane, un rifugiato politico fuggito della coscrizione obbligatoria in Eritrea che, come altre decine di migliaia di migranti, ha affrontato un viaggio disumano nel Mediterraneo, è stato incarcerato a Malta e poi è riuscito avventurosamente ad arrivare in Italia. Questo per dire che questo disegno di legge è nato prima di tutto fuori dalle Aule parlamentari. È nato sull'onda di una delle più grandi tragedie del mare, sulla quale speravo non si rinfocolassero in questo dibattito le polemiche, cosa che però puntualmente purtroppo è avvenuta. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti in discussione generale, a cominciare dal senatore Micheloni, che ha svolto un intervento appassionato e molto documentato, frutto anche dalla sua esperienza personale. La senatrice Albano ha giustamente auspicato coesione e solidarietà nell'affrontare questo provvedimento che non deve trasformarsi in un'inutile passerella di vanità politiche. E - aggiungo io - non deve essere neanche un modo per lavarsi la coscienza senza far seguire l'assunzione di responsabilità politica. Sento infine il dovere di rispondere agli interventi problematici che sono stati pronunciati, ossia a quei colleghi che legittimamente si sono detti scettici o contrari alle finalità di questo disegno di legge. Il senatore Liuzzi, ad esempio, ha parlato di pratiche farisaiche, di atteggiamento ipocrita della politica, di questa legge come uno specchietto per le allodole. Lo posso anche riconoscere: il rischio c'è, ma sta anche a noi, ad ognuno di noi, fare in modo che questa norma altamente simbolica diventi qualcosa di più e di diverso nella coscienza collettiva. L'unica cosa certa è che non possiamo limitarci ad assistere da spettatori a un fenomeno epocale come quello delle migrazioni dall'Africa e dal Medio Oriente. Al senatore Tosato, che ritiene questo disegno di legge e l'individuazione della data del 3 ottobre una mera operazione propagandistica, dico solo che, se anche fosse così, non sarebbe comunque nulla rispetto a chi la propaganda sugli immigrati la fa tutti i giorni dell'anno. signor Presidente: c'è bisogno in questo momento di coesione e di solidarietà e non deve essere questo provvedimento un modo per lavarsi la coscienza. Lo ripeto volentieri questo concetto. Ma dico no al populismo della paura, che parte dai problemi reali per passare a proposte tanto demagogiche quanto irrealistiche. Chiudere le frontiere e fare blocchi navali sono *slogan* che fanno sicuramente presa, ma la storia ha abbondantemente dimostrato che movimenti di popoli possano essere regolati ma non totalmente impediti e che non è stato ancora inventato un confine davvero invalicabile. Si dice poi di sospendere Schengen, ma è una prospettiva che sarebbe drammatica per la stessa esistenza dell'Unione europea e che per l'Italia si rivelerebbe disastrosa perché ci troveremmo nelle condizioni in cui si trova adesso la Grecia, dove sono bloccati decine di migliaia di rifugiati senza sbocco. Un'ipotesi del tutto realistica, visto che la chiusura delle frontiere macedoni sta per produrre un flusso verso l'Albania in direzione dell'Adriatico e quindi dell'Italia. Le immagini che le televisioni ci trasmettono dal campo profughi di Idomeni non sono degne di un'Europa civile. In questi giorni il confine tra Macedonia e Grecia è segnato dai mezzi blindati dell'esercito per fermare quella massa di migliaia di persone che proviene soprattutto dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan; persone che hanno viaggiato per mesi, hanno perso per strada figli, mogli e mariti, che sono state rinchiuse nei campi profughi in Turchia, che hanno raggiunto le coste e attraversato il mare con piccoli canotti a remi.

su un'intera generazione. Non ci sono mai state come oggi tante persone in fuga da persecuzioni politiche e guerre, molte delle quali cercano protezione proprio in Europa. Dobbiamo metterci nell'ordine di idee che, considerando le crisi in atto nei Paesi vicini, la situazione non cambierà nemmeno nei prossimi anni. Noi europei dobbiamo a noi stessi e al mondo una soluzione all'altezza della sfida che queste persone in cerca di aiuto rappresentano. Una cosa è emersa chiaramente: la risposta fornita finora non è all'altezza delle aspettative. L'Unione europea, a partire dal vertice di giovedì e venerdì prossimi, non può continuare a esitare e deve dimostrare prima di tutto di esistere. Ci deve essere uno *standard* di accoglienza di migranti che valga per ogni Stato membro dell'Unione e serve una politica di asilo europea. I profughi devono essere redistribuiti in maniera equa in tutta Europa. Una situazione come quella attuale, in cui pochi Stati membri devono gestire tutte le responsabilità dell'accoglienza, è insostenibile, di un sistema che fa gravare il peso in modo sbilanciato solo sui Paesi di confine. Abbiamo bisogno, dunque, di criteri vincolanti per una distribuzione dei rifugiati in base alla capacità degli Stati di gestirli.

a quello che sta avvenendo. Possiamo accoglierli tutti? Sicuramente no e per questo dobbiamo incoraggiare nuove iniziative politiche e misure per combattere le ragioni alla base dell'emigrazione dai Paesi del Medio Oriente e dall'Africa. La stabilizzazione della situazione di Stati che si stanno decomponendo e, poi, la creazione di reali prospettive economiche e sociali sono l'unica strada percorribile. Sembrano utopie (in effetti, in questo momento lo sono), ma se non si comincerà a ragionare e a operare fuori dalla logica emergenziale, l'Europa finirà sepolta sotto la propria impotenza. Signor Presidente, In alcuni interventi di ieri è stata messa sotto accusa l'operazione Mare nostrum, che è terminata il 1° novembre 2014. Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, migrazioni, nei primi quattro mesi del 2015, 900 persone sono morte nel canale di Sicilia. Nello stesso periodo del 2014, quando era in atto l'operazione Mare nostrum, i morti erano stati 96. Non solo, nei primi tre mesi del 2015, sono sbarcati 22.979 migranti contro i 20.899 del 2014. Si tratta in tutta evidenza di una cifra che smentisce un luogo comune molto diffuso, ossia che l'immigrazione era aumentata perché l'operazione Mare nostrum garantiva un passaggio sicuro ai migranti dal Nord Africa. Infine, nel primo mese dopo la fine dell'operazione, gli arrivi aumentarono del 485 per cento rispetto al novembre 2013, quando invece l'operazione Mare nostrum

ai precedenti storici delle migrazioni degli italiani verso l'estero. Si tratta di pagine di storia che l'Italia non ha adeguatamente valorizzato e che meritano di essere ricordate.

un nuovo rinvio alla Camera, una nuova navetta, sarebbero uno schiaffo in faccia ai promotori, che ci hanno così pressantemente chiesto che questo disegno di legge venisse approvato. Per questo chiedo al senatore D'Alì

Signor Presidente, quello che il Senato sta per approvare è un atto importante, come testimonia del resto la qualità degli interventi che ci sono stati. Si è detto che è un simbolo, ma io penso che la democrazia abbia bisogno di simboli e di punti di riferimento in cui riconoscersi e l'accoglienza è un simbolo di una democrazia aperta. Per questo è importante

di buonismo, né di pietà; non c'è alcuna rilassatezza dal punto di vista della capacità di controllo, ma, al contrario, questo testo testimonia consapevolezza, legalità e senso civico, tre aspetti che sono tra i pilastri delle nostre democrazie. Dall'accoglienza rispettosa della legge si misura il grado di civiltà delle Nazioni. Per questo è importante che nelle scuole e a partire da esse questa consapevolezza venga affrontata e diffusa. Rispetto a ciò che accade, la risposta sta nel controllo dei confini europei e non negli sbarramenti ai confini nazionali. Per questa ragione e per la qualità delle democrazie, Schengen deve vivere e non morire. Vorrei dire al senatore Liuzzi che ciò che ha affermato nel suo intervento, richiamando la necessità di una politica comune di accoglienza, è esattamente quello che si immagina anche con l'approvazione di questo testo di legge. Per cui davvero lo invito a ripensare e a sostenere in modo convinto questo provvedimento. Abbiamo bisogno di un'Europa politica e di un'Europa sociale. È giusto ripensare in chiave europea il Trattato di Dublino: anche questo aiuta a far vivere Schengen. Credo che questo sia appunto il tema che affronteremo anche oggi pomeriggio, con il Presidente del Consiglio, in attesa del nuovo appuntamento del Consiglio europeo sul grande tema del governo dei processi migratori. Credo che ci siano davvero tutte le condizioni perché, come sostenuto dal relatore, questo Parlamento a grandissima maggioranza possa dare un'ulteriore testimonianza della qualità del nostro sistema democratico.

si conviene sull'opportunità che questa giornata della memoria riguardi anche i temi dell'emigrazione italiana verso altri Paesi e poi, nella sostanza, al momento dell'approvazione degli emendamenti, non si consente che ciò accada, per motivi di urgenza. Non so chi abbia preso impegni anche nei tempi. L'impegno che qualcuno ha preso con un'associazione era quello di portare la legge in Parlamento; ma il Parlamento poi è sovrano nelle sue determinazioni e ha l'obbligo di ricondurre il tema ad un equilibrio complessivo, nei confronti soprattutto dei giovani. Il Ministro della pubblica istruzione, a seguito di questa norma,

dell'immigrazione verso il nostro Paese e non sarà l'occasione per poter ricordare ai nostri giovani un fenomeno straordinariamente importante nella nostra storia, che è quello dell'emigrazione italiana. Credo che abbiamo il dovere di reggere con equilibrio tutte le questioni, al di là degli impegni che qualcuno può avere preso al di fuori di questa Aula. L'Assemblea è tale perché deve, con assoluto equilibrio, esaminare tutte le vicende. Istituire una giornata non è

dia un indirizzo celebrativo e pedagogico nelle nostre scuole riguardo ai temi dell'immigrazione e trascuri i temi della grande epopea dell'emigrazione italiana,

Lo abbiamo affrontato nel Comitato già nel 2007 e lo abbiamo ripreso ultimamente con il ministro Giannini. C'è una discussione in corso su questo tema.

è molto utile per comprendere l'immigrazione nel nostro Paese. I nostri connazionali sono emigrati secondo le regole di un ingresso legale negli Stati Uniti d'America e negli altri Paesi

serve invece a garantire un approfondimento culturale necessario nelle scuole e in tutti gli organismi già deputati a tale scopo.

nei giorni scorsi si è ricordato il venticinquesimo anniversario del primo grande esodo degli albanesi sulle coste pugliesi. Tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo del 1991 il Basso Adriatico e il canale d'Otranto registrarono il passaggio di circa 27.000 albanesi che, fuggiti dal regime ormai vacillante di Ramiz Alia (erede del dittatore Enver Hoxha), cercavano nel nostro Paese la loro terra promessa. L'Italia scoprì in quei giorni di essere diventata terra di immigrazione. I pugliesi nei decenni precedenti avevano abbandonato la propria terra e le loro famiglie alla volta delle città nel Nord dell'Italia e dell'Europa. Prima

Signor Presidente, stavo dicendo che quei pugliesi, quegli stessi cittadini meridionali, che erano stati protagonisti di pagine anche tristi di emigrazione, invece in quegli anni e nel 1991 scoprirono di trovarsi di fronte a un altro fenomeno, che era quello dell'immigrazione sulle nostre coste, dando prova delle proprie capacità di accoglienza che furono apprezzate in Italia, in Europa e in tutto il mondo occidentale. Se ricordate, addirittura ci fu chi propose il premio Nobel per le popolazioni pugliesi. Come dicevo, il nostro Paese, da sempre terra di migrazione, dovette cimentarsi con un fenomeno totalmente nuovo. Il Governo, il Parlamento, le nostre classi dirigenti furono quasi costrette dagli eventi di quel 1991 a dover organizzare un sistema di accoglienza e gestione dei profughi e dei clandestini fino a quel momento mai predisposto. Solo qualche mese prima era stata approvata dal Parlamento la legge n. 39 del 1990, la legge Martelli, con la quale si cercò di regolamentare un fenomeno inedito, rispetto al quale il nostro Stato, nelle prime fasi, non diede una gran prova di efficienza. non rammenta il successivo episodio dell'8 agosto 1991, l'arrivo della nave Vlora nel porto di Bari e l'imbarazzante scenario dello Stadio della Vittoria? Questo è a dimostrazione di una Nazione e di un Governo che non avevano ancora capito di fronte a a quale scenario e a quale fenomeno si trovavano, che dovevano essere per forza gestiti. Sono trascorsi venticinque anni e oggi, in quest'Aula, ci troviamo ad esaminare e ad approvare il disegno di legge per l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. L'intento di tale iniziativa è certamente nobile. Non si può non ricordare che in questi venticinque anni i nostri mari e le nostre coste hanno registrato eventi tragici e luttuosi come quello del 3 ottobre 2013 - già ricordato - a a largo di Lampedusa, con 366 vittime e 20 dispersi, o come quello del 18 aprile 2015, nel Canale di Sicilia, con oltre 700 vittime. Si potrebbe, quindi, considerare la *ratio* del presente disegno di legge nell'intento di rendere sempre vivo nelle nostre comunità il ricordo di quelle e altre tragedie legate agli esodi dei migranti di tutta l'area mediterranea,

Tuttavia, non si possono non considerare, anche in questa occasione, tutti i problemi irrisolti e le questioni ancora aperte riguardo alla gestione dei flussi migratori e all'organizzazione dell'accoglienza. nel quarto di secolo appena trascorso, non sempre ha affrontato questo problema nel modo migliore, garantendo le soluzioni più idonee agli stessi profughi e ai propri cittadini. Lo spontaneismo che contraddistinse quella prima fase del 1991 è rimasto la cifra della macchina dell'accoglienza italiana, con gli inevitabili effetti collaterali. Dopo la citata legge Martelli, si sono succedute le leggi Turco-Napolitano e Bossi-Fini, ma i risultati concreti sono stati invero esigui e insoddisfacenti. Contemporaneamente l'Italia e, in particolare, i Governi degli ultimi anni non sono riusciti a coinvolgere appieno l'Europa, chiedendo ai Paesi membri una maggiore solidarietà e vicinanza per la soluzione di un problema divenuto ormai cronico, che non può riguardare solo noi. Proprio in queste ore si registra l'ennesimo *flop* dell'Unione europea; l'accordo con la Turchia stenta ad essere concluso; né, d'altronde, si riesce a sensibilizzare i Paesi nel Nord Europa sulla necessaria rivisitazione del regolamento di Dublino. Sono questi i giorni delle immagini eloquenti e raccapriccianti del campo profughi di Idomeni, del filo spinato alla frontiera macedone. Ci interroghiamo smarriti sul possibile perverso effetto domino di profughi che, dai Balcani, potranno indirizzarsi nuovamente verso il basso-adriatico e l'alto-ionio, andando ad interessare di nuovo Puglia e Calabria ionica. Ebbene, di fronte a questo scenario preoccupante e angosciante, il presente disegno di legge non ha altro effetto che quello di un banale placebo. Servirà sicuramente a diffondere una maggiore sensibilizzazione nelle nostre comunità e tra i nostri studenti, ma contemporaneamente rischia di sviare la nostra attenzione dalle questioni fondamentali tutt'ora irrisolte, cui facevo cenno prima,

Qual è la qualità del nostro sistema di accoglienza? Qual è l'affidabilità del nostro sistema di pubblica sicurezza nella gestione dei flussi? Perché non si riesce ad organizzare un sistema efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati? E potrei continuare. Ma prima di concludere, un pensiero doveroso va agli operatori delle Forze armate, della Marina militare, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, che hanno affrontato, spesso nelle condizioni più estreme, i momenti più difficili dell'accoglienza, risolvendo nei limiti del possibile, a volte anche dell'impossibile, le situazioni più disperate. Ad essi non può non andare il nostro sentito ringraziamento e la nostra totale vicinanza. Anch'essi meriterebbero riconoscimenti formali per la loro attività. Altro che giornate nazionali, ormai sin troppo inflazionate. Anche per questi motivi e per le ragioni evidenziate all'inizio del mio intervento, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti non potrà esprimere il proprio voto favorevole, limitandosi a un voto di astensione, perché altro non si può fare di fronte alle questioni irrisolte prima accennate, e che solo qualche giorno fa il senatore D'Ambrosio Lettieri aveva riproposto chiedendo

ovvero l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Ieri ho sentito parlare di tutto, soprattutto e solo di immigrazione: di Giornata della memoria ho sentito parlare ho sentito parlare poco. Cosa voglio dire? Innanzi tutto, l'istituzione di una Giornata nazionale è assolutamente inutile, perché ritengo completamente inflazionata la materia. Dovrebbe essere considerato offensivo istituire un'altra giornata quando ci si riferisce a delle vittime, a dei poveretti morti in mare. Lo dico perché - per chi non lo sapesse - le nostre giornate più o meno ufficiali dedicate a qualcosa sono 253: 253: brilliamo per la giornata dedicata al gatto; alla difesa della rana, alla lentezza, agli UFO, e non può mancare la giornata degli angeli custodi. E probabilmente avremmo bisogno anche qui di angeli custodi per evitare di istituire l'ennesima Con quelle ufficiali, partendo proprio da oggi e arrivando fino al 2 giugno, praticamente ce n'è una ogni due o tre giorni. Anche stamattina strage di via Fani, dove sono sempre presenti ogni tre giorni il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, il Capo di Stato maggiore. Mi chiedo se, in un momento in cui l'ISIS minaccia i Paesi occidentali, forse non sarebbe il caso di mandarne uno a rappresentare il Paese. Se dovesse infatti intervenire un attacco in quell'occasione, tutti sarebbero alla giornata di commemorazione e nessuno difenderebbe i patri confini.

le coste da cui potrebbe riaprirsi la migrazione attraverso il Canale di Otranto e noi, differentemente da tutto il resto del mondo, andiamo a istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. venite qui perché la strada giusta è quella del Canale di Otranto. D'altra parte, credo sia la politica - è sempre stata sottesa, dal Governo Monti a quelli di Letta e Renzi - ad aver portato a questi risultati, perché ho sentito numeri numeri che possono essere ampiamente contraddetti anche da parte del relatore, senatore Mazzoni. Io ho visto solo una cosa: fra Mare nostrum, Triton e Poseidon abbiamo portato a casa,

35 volte il numero dei morti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi, non veniteci a dire che queste operazioni hanno ridotto quella mortalità, perché è accaduto esattamente il contrario. Mi spiace di vedere, poi, anche una certa ipocrisia perché noi, adesso, facciamo una corsa e addirittura non si accettano modifiche al testo perché bisogna essere pronti almeno per il 3 ottobre dell'anno prossimo per i morti di Lampedusa.

per cento vorrebbe chiudere di nuovo e subito tutti i confini nazionali. Si tratta di due numeri sorprendenti nel Paese che, solo qualche anno fa, credeva ciecamente nelle magnifiche sorti e progressive dell'unificazione del vecchio continente.

un tempo eravamo quelli che all'Europa credevano più di tutti, quasi in un modo romantico, sentimentale: eravamo innamorati dell'Europa, ma adesso la gente capisce che il governo europeo non c'è. C'è la Germania che cerca di essere umanitaria, c'è la Francia che decide di essere rigorosa, c'è una Commissione europea che stabilisce delle regole per l'accoglienza dei rifugiati, ma poi nessun Paese le rispetta. La sfiducia nell'Europa e la voglia di rimettere le guardie alle frontiere portano alla luce un dato interessantissimo, la terza cifra che non ti aspetti. per cento dei simpatizzanti del Partito Democratico che si schiera contro Shengen rivuole i confini. Certo, è un numero inferiore a quello dei leghisti e dei forzisti, ma rivuole i confini. Come si spiega?

Certo, un peso hanno i *media* che dipingono ogni giorno un'Europa nel caos. Ma la cruda verità è che le stesse persone che si sforzano di dimostrare che quello degli immigrati non è un problema - parlo degli italiani di sinistra - in realtà pensano che lo sia. Non hanno il timore di perdere il posto di lavoro, ma sentono l'allarme per una nuova criminalità che, purtroppo, i dati reali confermano e c'è la paura che gli immigrati siano loro concorrenti nel *welfare*, nell'assegnazione delle case - per esempio nelle file al pronto soccorso. La sinistra ha risolto il problema non affrontandolo: semplicemente non ne ha parlato. Ha dato tutta la colpa all'Europa e stop. Queste cose le scrivono «la Repubblica» e credo illustri professori. Ma è finito il tempo di dare la colpa all'Europa, perché in questo momento ha assunto un atteggiamento completamento diverso dal nostro: sta reagendo. Mentre noi siamo qui a parlare di queste cose,

Come li chiamate voi se non respingimenti? Solo che, quando di respingimenti e di rimpatri ne parlava la Lega, eravamo dei razzisti, mentre oggi sono razzisti la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, l'Austria. Questi sono i Paesi razzisti o siamo noi dei matti?

e della memoria dei migranti, evidentemente stiamo parlando dei clandestini e non di coloro che vengono qui sfuggendo alle guerre. Ma quando gli altri Paesi mettono dei limiti numerici oppure bloccano le frontiere, noi ci inventiamo di andare a prenderli sotto le coste libiche; ci siamo inventati l'abolizione del reato di immigrazione clandestina; qualcuno cerca di far passare anche l'espansione della cittadinanza applicando lo *ius soli,* ovvero lo *ius culturae*. Ieri ho sentito qualcuno dire che erano cittadini francesi e belgi quelli che hanno fatto gli attentati a Parigi. Sono diventati cittadini europei, francesi e belgi, grazie allo *ius soli*, e noi in questo momento cerchiamo di introdurlo a casa nostra. Non solo e non basta, perché ci si è inventati lo *ius culturae*, che rappresenta veramente il rischio di qualcosa che viene meno nostra identità e della sicurezza a casa nostra, perché noi intendiamo dare la cittadinanza non a coloro che sono venuti nel nostro Paese entro una certa età e hanno studiato: la diamo anche a chi non ha conseguito un titolo di studio, come nel caso della formazione professionale. Quindi, sarà

Mi fa rabbrividire l'idea che noi siamo qui a far questo, mentre Renzi sarà a dialogare in sede europea con un Paese come la Turchia che va con l'ISIS, che si permette di chiudere i giornali dell'opposizione e di controllare completamente l'informazione: sarà a dialogare con dei ricattatori che chiedono dei soldi

per cosa? Per tenerli a casa loro e farli morire di fame e di freddo? Non vi sentite un po' ipocriti nel girarvi dall'altra parte e stare qui oggi a festeggiare? Oggi c'è solo da festeggiare una sconfitta: la sconfitta di tutta la politica migratoria e immigratoria dell'Europa. *(Applausi

dell'Italia, dell'Europa e anche della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. È dunque un momento importante. È importante anche il giorno scelto, il 3 ottobre,

garantisce allo straniero il diritto di asilo in Italia, e non per le persecuzioni che subisce nel suo Paese, ma per il fatto che nel suo Paese non gli vengono garantite le stesse libertà democratiche che ha che ha un italiano, che ha una persona che vive in Italia. Quindi, prendiamo come riferimento e come modello - ed è giusto che sia così - le nostre libertà democratiche e cerchiamo di darle a tutti quelli che, non potendole avere nel loro Paese,

D'altra parte, per noi italiani, una celebrazione di una giornata, riferita a persone che, appunto, hanno rischiato la vita e, in alcuni casi, l'hanno persa per venire da noi, è in fondo un riconoscimento di ciò che è diventata l'Italia: un modello per i Paesi del mondo, e non solo di natura economica

e della nostra migrazione, l'Argentina, già nel 1995 ha istituito il 3 giugno come Giornata dell'immigrante italiano.

il senatore Calderoli

agli approcci non positivi da parte della Comunità europea che si sono registrati nel

questo stia comportando, anche per quanto riguarda Schengen. Vi è quindi uno sviluppo nelle ultime settimane, nell'approccio alla questione dei migranti in Europa, che si sta materializzando solo nelle politiche della chiusura, del respingimento e nella fredda indifferenza verso la vita di milioni di persone. I drammi che si succedono e i morti annegati

dalle parole attraverso cui il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si è espresso proprio qualche giorno fa, a conclusione della riunione dei Capi di Stato e di Governo europei con la Turchia il 7 marzo.

quindi un incardinamento vero di serie politiche di accoglienza e dell'immigrazione e anche alcuni punti molto chiari sull'agenda europea,

di gestione dei flussi migratori da un Paese all'altro. Si continua a non comprendere che ci troviamo di fronte a un esodo di massa e il fatto che l'Europa possa nascondersi dietro le politiche di respingimento e di chiusura delle frontiere è un'idea che non solo respingiamo dal punto di vista politico, etico e valoriale, ma è anche irrealistica, perché non vuole assolutamente fare i conti in modo chiaro e preciso con quello che è davanti a noi. Il fenomeno dell'immigrazione è strutturale. Oggi

che voglio qui richiamare con forza, per un motivo molto semplice: una delle questioni che facciamo finta di non vedere è che in Italia e in Europa non c'è più modo di entrare in modo legale. Quali sono i canali? abbiamo parlato varie volte di canali umanitari e di organizzare in modo serio l'ingresso in Europa e nel nostro Paese, ma su questo non ci si vuole confrontare e l'Europa mostra una chiusura totale. totale. Qui ancora si richiamano i clandestini, ma io rivolgo a tutti noi una domanda: quali sono oggi i canali di ingresso legale nel nostro Paese e in Europa?

gli immigrati entrati in modo legale, a dimostrazione che si può costruire con serietà una politica di ingressi attraverso i canali umanitari.

solo richiamare a tutti noi i valori dell'accoglienza. Una società come la nostra non può non misurarsi con questo. Serve anche per assumerci degli impegni

è inutile che facciamo finta di niente - ci dovremo misurare per molti anni ancora. Per tutti questi motivi esprimiamo un voto favorevole al disegno di legge in

voterò. Si apre una questione di fondo politica, morale e culturale che è stata sottolineata ieri in maniera esemplare dal collega Micheloni. In un bellissimo intervento egli ha infatti sottolineato come le tragedie dell'immigrazione e delle persone che perdono la vita in mare - di questo si tratta - abbiano connotato tutta la fase dell'emigrazione italiana verso l'estero. Ha citato circa sei naufragi in cui dai 200 ai 500 connazionali hanno perso la vita mentre migravano all'estero e ha documentato un fenomeno migratorio che ha interessato 60 milioni di italiani andati all'estero e che oggi interessa milioni di persone che cercano salvezza da situazioni di guerra o per ragioni economiche.

agli immigrati, a quelli che hanno perso la vita in mare venendo in Italia. Questo peggiora di gran lunga la situazione. Vorrei chiedere ai colleghi, anche sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, che differenza esiste tra un emigrato italiano che andava in giro per il mondo e ha perso la vita per mare e un immigrato che viene in Italia e perde la vita per mare.

questo è il luogo in cui collocare, giustamente, il ricordo e la prospettiva storica del fenomeno, se vogliamo dire ai giovani che quello che oggi tocca alle persone che vengono dall'Africa o dall'Asia, un giorno era toccato ai nostri emigranti, che per necessità dovevano andare all'estero.

moralmente e politicamente indifendibile, perché non riconosce questa parità di condizioni, che è essenziale. Naturalmente ciò fa nascere

non ci siano grandi controindicazioni nel condividere un disegno di legge che ha degli obiettivi assolutamente meritori.

che è molto più semplice rispetto agli argomenti, sia pur valoriali, che sono stati esposti oggi da chi mette in discussione il provvedimento. Ritengo che, come è stato detto, la decisione di ricordare un dramma umano, che ha riguardato migliaia e migliaia di persone persone morte in mare per sfuggire alla povertà, alle persecuzioni, alla paura e all'odio, sia cosa buona e giusta.

Non possiamo tradire quello che stiamo vivendo, ma dobbiamo renderlo imperituro nei ricordi e nella storia. D'altronde si tratta di un disegno di legge che non prevede una celebrazione, non prevede feste, non prevede feste, interruzioni lavorative o interruzioni delle lezioni scolastiche; prevede soltanto che, sulla base delle direttive ministeriali, quel giorno le istituzioni, soprattutto quelle scolastiche, si muovano si adoperino per ricordare questa triste vicenda umana. Non siamo qui, signor Presidente, per lavarci la coscienza, ma per riempire le coscienze di ognuno di noi e per sensibilizzare la coscienza

questa è un'occasione per coinvolgere molti Stati dell'Unione europea che fino ad ora sono stati sordi, riluttanti e non ci hanno aiutato e che soltanto ora hanno preso coscienza di quanto questo fenomeno sia pericoloso per la nostra integrità sociale. I dati che ci forniscono i nostri istituti sono veramente terribili. Le tristi vicende degli ultimi tempi hanno indotto i Paesi europei ad un atteggiamento di maggior risolutezza nell'affrontare questo fenomeno è stato predisposto un meccanismo di ricollocazione dei migranti, che però stenta ad avviarsi nella maniera L'Italia sta facendo la propria parte nel costruire le strutture di prima identificazione e nella rilevazione delle impronte digitali dei migranti e nell'accoglienza, ma ancora siamo assolutamente in ritardo, infatti

c'è bisogno che l'Europa faccia di più. Infatti, secondo gli ultimi dati della Commissione europea, sui 160.000 posti che avrebbero dovuto essere messi a disposizione dagli altri Stati dell'Unione europea nel meccanismo di ricollocazione, attualmente sono stati forniti posti solo per 6.900 migranti. migranti. Dalle cifre richiamate capiamo quindi che l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione rappresenta un monito per una profonda riflessione su un fenomeno che ancora oggi assume proporzioni difficilmente governabili, ma che solamente attraverso l'unione di tutti i Paesi europei sarà possibile affrontare nel rispetto della dignità della vita umana e del diritto alla

Ipocrisia, falsità e complicità: sono queste le parole che mi vengono in mente quando sento parlare di istituire una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Potevamo impiegare questo tempo per tentare di risolvere i problemi legati alla gestione dell'accoglienza degli immigrati e invece il tempo lo stiamo perdendo per istituire una giornata della memoria che non risolve niente e non serve ai cittadini; non neanche alle vittime e ai familiari delle vittime o ai loro parenti e amici. Serve solo ad imbastire il vostro teatrino dell'ipocrisia: da una parte ci sono quelli che «immigrati a casa, sempre e comunque» (anche se una casa non ce l'hanno più, perché gliel'abbiamo distrutta); dall'altra quelli che pensano di lavarsi la coscienza con le giornate della memoria. Fatevela da soli questa legge. Noi non siamo complici di chi blocca il Parlamento a fare cose inutili e poi si presenta in tv a fare la parte degli statisti. Questa è una legge alla memoria dei disperati, ma mangiate sulle cooperative che quei disperati cercano di accogliere. per celebrare la memoria delle vittime dell'immigrazione, quando Alfano è ancora il ministro dell'interno, quando le cooperative, da destra a sinistra, mangiano sugli immigrati. È solo un modo per pulirvi la coscienza con il sangue dei disperati, di quei disperati che voi per primi avete contribuito a rendere tali bombardando i loro Paesi. Lo fate per nascondere Mafia Capitale, lo fate per nascondere le vergogne dei CARA e dei CIE, sui quali avete speculato, elettoralmente e non solo. L'ipocrisia della propaganda riguarda anche colleghi della Lega, che dicono «40 euro a immigrato» quando quei soldi sappiamo che poi se li fregano le cooperative (o di destra o di sinistra, non importa). È vergognoso che il Parlamento della Repubblica, al posto di una legge sul conflitto di interessi, di una legge sull'anticorruzione, di una legge per affrontare il problema delle imprese, dove gli imprenditori e gli operai si ammazzano, di un reddito di cittadinanza, che possa creare quelle condizioni di vita tali da rendere questo Paese più accogliente, utilizzi il tempo per l'istituzione di una giornata della memoria. Abbiamo perso due giorni della settimana. Ieri un altro pomeriggio inutile, di discussione inutile: diciamolo. Un dibattito ridicolo in questi anni su come risolvere il problema dell'immigrazione, su come contrastarla, su chi se ne approfitta di più, su chi è più sensibile alle vittime e chi meno. Si affronta l'immigrazione come un problema da combattere per qualcuno e una manna dal cielo per qualcun altro; una bandiera elettorale su cui far convergere i propri elettori, i buonisti da una parte e i cattivi dall'altra, per etichettare quelli di una parte e quelli dell'altra, e ciascuno fa la sua parte. Dove stavate durante il semestre europeo, quando dicevate che avreste risolto il problema dell'immigrazione? Così lo risolvete, con la giornata in memoria delle vittime? L'ipocrisia perbenista uccide questo Paese. Più dei corrotti e più dei ladri, il dramma sono i disonesti intellettuali, quelli che poi prenderanno voti dicendo che hanno affrontato il problema dell'immigrazione con inutili leggi come questa. L'Italia è travolta dalla corruzione, dai conflitti d'interesse, dalla burocrazia, dalle *lobby*. Non passa giorno che non arrestino qualcuno di voi per mazzette, tangenti, abuso d'ufficio e chi più ne ha più ne metta. C'è un Paese dove appena piove crollano strade, ponti e case. Ci sono cittadini che si ammazzano perché perdono il lavoro, la casa e non hanno più un reddito. Ci sono scuole in cui i ragazzi sono accampati. E voi sprecate tempo e soldi pubblici ad istituire giornate della memoria. Servono le leggi; serve il sequestro di chi ci campa, di chi lucra sugli immigrati, il sequestro di quei terreni dove gli immigrati lavorano in nero e ci lavorano grazie ad accordi politici di destra e di sinistra. Serve trasparenza in quelle cooperative che mangiano sul disastro dell'immigrazione e sono cooperative cielline, falsamente cattoliche, e cooperative rosse, falsamente comuniste. Oggi stiamo parlando dell'istituzione di una giornata della memoria e non di soluzioni alla immigrazione e ai morti in mare; quelli li risolviamo se iniziamo a rispettare ciò che anche voi avete votato alla Camera nella mozione del 18 dicembre scorso, in cui il Movimento 5 Stelle ha presentato sette punti chiari

Il tema dell'immigrazione deve rimanere irrisolto per permettervi di raccattare voti in campagna elettorale, da una parte e dall'altra. Se si affrontasse seriamente, molti di voi perderebbero la poltrona. Per questo ci asterremo. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia non voterà favorevolmente questo provvedimento. Mi rivolgo anche al collega Crimi: non è scandaloso che il Parlamento occupi due sedute per esitare un disegno di legge su una giornata della memoria; è scandaloso che ciò accada su un *input* esterno per un accordo fuori dal Parlamento e che lo stesso Parlamento, pur riconoscendo l'opportunità di doverlo modificare, non riesca a farlo. Così è stato detto dal relatore. questa è una Giornata della memoria dimezzata. Noi vogliamo che i nostri giovani abbiano una parziale visione del fenomeno dell'immigrazione, fenomeno storico fenomeno storico assolutamente collegato soprattutto alla nostra storia (e parlo, come ho detto in discussione generale, da siciliano), e si vuole pure ostentatamente evitare che che in un unico contesto venga decisa una cosa che poteva essere decisa serenamente e - vorrei dire anche - quasi con l'accordo di tutti. La solita logica dei numeri che prevale sulla logica del ragionamento, della razionalità, sulla logica di ciò che sarebbe più corretto fare. Ma a forza di andare avanti con questo sistema

sia quelli originariamente scelti dal popolo italiano sia quelli occasionalmente catturati nell'ambito dei corridoi e dei palazzi parlamentari. Prima o poi questo vi capiterà, e allora questo vostro atteggiamento di assoluta chiusura alla possibilità di un ragionamento un po' più complessivo

complessivo dell'educazione da dare ai nostri giovani. Volete che tutto sia ricondotto in quest'ambito: non avrete il nostro voto favorevole.

Le ragioni di un voto favorevole sono state già espresse negli interventi assolutamente

dunque gli argomenti sono stati svolti pienamente in quest'Aula. Colgo piuttosto questa occasione per esprimere il mio pensiero sulle cose che sono state dette in dichiarazione di voto, che non mi possono lasciare indifferente per la loro aggressività e perché mi sembrano assolutamente sbagliati gli argomenti usati e inopportuni gli atteggiamenti adottati da alcuni Gruppi politici. Voglio ricordare a tutti che questa doveva e vuole essere una giornata contro l'indifferenza; una giornata in cui l'Italia (quella parlamentare, l'Italia del Governo, l'Italia delle istituzioni), anche a seguito dello stimolo dato dal Comitato 3 ottobre - che, partendo da Lampedusa, ha raccolto 30.000 firme - vuole vuole dire una cosa molto semplice: che quei 368 morti in mare non ci lasciano indifferenti. Certo, di morti in mare prima e dopo ce ne sono stati tanti altri, quindi noi cogliamo quello che è stato un evento simbolo, nell'accezione che del simbolo ha dato il collega Manconi. Siamo consapevoli che gli immigrati morti in mare non finiscono il 3 ottobre

che sono stati raccolti in mare e sono stati distribuiti per essere seppelliti in tutta Italia, è un dovere ed è anche l'occasione per un Paese come il nostro per dimostrare, come ha detto il sottosegretario Pizzetti, il grado di civiltà del Paese stesso. Questa mattina non stiamo discutendo di politica dell'immigrazione

il provvedimento successivo, Triton, che è ispirato agli stessi principi, ma tante altre cose sono accadute anche fuori dalle istituzioni elette. Penso, ad esempio, alla condanna a trent'anni - che ha retto nelle sue argomentazioni

ed emigrati; stiamo parlando del dovere di uno Stato come il nostro che, rispetto ad un'Europa civile,

anche come Paese oltre che come soggetti, di guardare verso gli altri. In questo momento non stiamo parlando di emigrazione ma stiamo guardando, con la sensibilità di un Paese che conosce l'emigrazione e la sua sofferenza, all'immigrazione di altri che, lasciando miseria e guerra, si sono accostati al nostro Paese. Dov'è allora la contraddizione? Io ho approfittato dell'ostinata volontà del collega D'Alì di modificare il testo per cercare di dire una cosa molto importante c'è una scelta politica di fondo. Non è vero che ci siamo dimenticati degli emigrati. Nessuno può dimenticarsi degli emigrati e non è un caso che il Gruppo del PD abbia affidato una delle dichiarazioni più importanti ad un collega che sull'emigrazione ha costruito la sua storia sua storia e la storia della sua famiglia. Essere consapevoli della sofferenza che provoca l'emigrazione ci rende più ricchi, più sensibili, più accoglienti. Ci consente, cioè, di avere quel grado di civiltà e di consapevolezza che, davanti all'episodio di Lampedusa, non solo il nostro cuore e la nostra sensibilità ma ci fa considerare quello come un momento fondante della civiltà di un Paese. Ieri, per conto del Senato, ho accolto alcuni studenti per discutere con loro della Giornata del 17 marzo

hanno senso le giornate della memoria? Ha senso questa Giornata? Ha senso la Giornata dell'Unità nazionale? Ha senso la Giornata, di cui parleremo subito dopo, in ricordo delle vittime di mafia? E mi sono sentita dire da tanti di quei ragazzi: «Sì, ha senso, perché noi la nostra storia spesso non la conosciamo, perché i fatti diventano fatti di cronaca e di storia tanti anni dopo, e noi delle cose che succedono in Italia sappiamo poco perché nelle scuole ci avete tolto anche la possibilità di approfondire». Queste giornate indirizzate all'approfondimento servono allora a questo: a trasmettere il senso di una memoria che ci rende popolo che ci rende popolo più civile, soprattutto perché accogliente, perché sofferente, perché capace di apprezzare e di capire sino in fondo le sofferenze degli altri. Quelle persone non vanno dimenticate, anche perché la nostra politica ne deve tenere conto e perché l'educazione dei nostri studenti non può prescindere dal ricordo in queste Giornate.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 aprile. Questa mattina, subito dopo la definizione del calendario dei lavori, si passerà all'esame del disegno di legge sulla giornata della memoria delle vittime delle mafie, fino alle ore 14. Ove non conclusa, la discussione generale su tale provvedimento proseguirà questa sera, dopo il voto sulle risoluzioni concernenti le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo. Nella seduta antimeridiana di domani, oltre al seguito del disegno di legge sulle vittime delle mafie, inizierà l'esame del disegno di legge sul terzo settore. Al fine di concludere la discussione generale, per la seduta antimeridiana di domani non è previsto orario di chiusura. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 12 di domani. Nella seduta di *question time* di domani pomeriggio il Ministro della salute risponderà a quesiti su aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e prevenzione vaccinale e profilassi. L'esame degli emendamenti al disegno di legge sul terzo settore inizierà a partire dalle ore 15 di martedì 22 marzo, con prosieguo fino al voto finale del provvedimento nella seduta unica di mercoledì 23. Entrambe le sedute della prossima settimana non prevedono orario di chiusura. Dopo le festività pasquali, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalle ore 10,30 di mercoledì 30 marzo. Il calendario di quella settimana prevede la discussione delle relazioni della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nonché delle mozioni sulla sottrazione internazionale di minori, su Boko Haram, sulla stabilizzazione degli *ecobonus*, sulla privatizzazione delle ferrovie e sul sindacato ispettivo. Sarà inoltre esaminato, ove concluso dalla Commissione, il disegno di legge sul reato di negazionismo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Nel pomeriggio di giovedì 31 marzo si svolgerà il *question time*con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nella settimana dal 5 al 7 aprile saranno discussi il decreto-legge sulla riforma delle banche di credito cooperativo, in corso di esame presso la Camera dei deputati, nonché, ove conclusi dalle Commissioni competenti, i disegni di legge sulle agenzie ambientali e sulla concorrenza. Infine, il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di cinema. Durante le discussioni generali in Aula le Commissioni potranno convocarsi,

continuiamo a non comprendere per quale motivo - è una questione che dura da molto tempo - non si voglia procedere nel senso di ratificare una decisione di un'amministrazione e di una comunità che si è espressa secondo le norme. La questione è stata anche affrontata nella Conferenza della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ripropongo con forza la questione dei disegni di legge delle opposizioni. che impegna il Governo e tutti noi ai tempi previsti dal nostro Regolamento per rispondere a tutti gli atti di sindacato ispettivo, che è una questione molto grave qui al Senato perché il Governo perché il Governo non risponde praticamente mai. Per di più, vorrei ricordare sempre ai colleghi senatori che il nostro *question time* non è come quello della Camera perché qui i Ministri rispondono soltanto alle domande a cui fa piacere rispondere e non a quelle che noi liberamente poniamo. vorremmo sapere come possiamo svolgere fino in fondo la nostra funzione anche rispetto ai cittadini che rappresentiamo. La stessa questione riguarda i disegni di legge dell'opposizione, che abbiamo posto varie volte.

Presidente Napolitano, ora senatore a vita, secondo cui l'Assemblea dovrebbe lavorare dal lunedì al venerdì, rilevo che nel calendario approvato per le prossime settimane,

il Senato "chiude" da giovedì 24 a martedì 29. Sono ben sei giorni, in cui l'Assemblea decide di interrompere i propri

chiedo di calendarizzare la mozione sull'ISEE, in quanto, a seguito di varie sentenze del TAR,

non può essere inserito l'assegno di accompagnamento dei disabili. Dato che tanti senatori in questa Assemblea sono molto vicini ai

tutte le prestazioni assistenziali e vengano rimborsati tutti quei cittadini italiani e quelle famiglie che a fatica riescono a vivere. quantomeno a loro non tolto un diritto che deve essere riconosciuto, acquisito e che non può essere ricompreso all'interno del calcolo dell'ISEE. il Governo abbia qualche difficoltà nell'inserire una previsione del genere, dato che nel disegno di legge sulla povertà, in questo momento in discussione alla Camera, si pensa di andare a collegare al calcolo dell'ISEE le pensioni di reversibilità o gli assegni sociali o l'integrazione al minimo. Quindi, le intenzioni sono sempre quelle di andare a colpire i più deboli e i più poveri. È dunque arrivato il momento che quest'Assemblea dimostri davvero - non a parole, non quando si va a parlare con un singolo cittadino, non nei TG, non nelle trasmissioni televisive, ma con i fatti

dal Governo che ha suggerito a entrambi, con un accordo, di portare avanti questa scelta scellerata. Ciò può solo dimostrare la volontà di parlare di autonomia, di federalismo, di temi che non sono assolutamente più nel DNA di certi partiti.

un provvedimento legittimamente votato. Se per voi il *referendum* ha ancora un valore, vi chiedo di rispettarlo e di calendarizzare nuovamente il provvedimento

nasce un certo fastidio in molti partiti che sono rappresentati in quest'Aula e in Parlamento. Le parole *referendum* e sovranità popolare danno fastidio. Dà fastidio - ad esempio - rispettare il *referendum* sull'acqua pubblica, come abbiamo visto qualche giorno fa. Dà fastidio: 26 milioni di italiani si sono espressi per l'acqua pubblica, ma dà fastidio votare una legge che stabilisce che l'acqua non possa essere privatizzata.

questo caso parliamo di un*referendum* di minori dimensioni, che riguarda un Comune, anche piccolo, del Veneto. Ma rispetto a questo si erano espresse favorevolmente anche le Province di Belluno e di Udine e si erano espressi favorevolmente anche i Consigli regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Giulia. Qualcuno potrebbe sostenere, nel merito del provvedimento, che mancano che mancano i presupposti di tipo geografico, storico, culturale, economico, religioso, politico o linguistico. Ebbene, non è vera alcuna di queste

grande percentuale di consenso rispetto all'unione con il Friuli-Venezia Giulia. Chiaramente la mia richiesta è prevedibile. Il Movimento 5 Stelle

attesa media. Invece, mio malgrado, prendo atto della inqualificabile volontà della maggioranza di posticipare la trattazione dell'argomento concernente il trasferimento del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia. Anzi, mi pare di poter dire che prendo atto della volontà del Partito Democratico di procrastinare *sine die* la trattazione dell'argomento, evitando in ogni modo la possibilità di approdo in con ciò esprimendo una posizione politica incapace di dare le dovute risposte, positive o negative che siano, alle popolazioni interessate; con ciò esprimendo, tra l'altro, una posizione politica non trasparente e - a mio avviso - decisamente arrogante. Sarebbe stato meglio che il Partito Democratico non avesse calendarizzato affatto questo disegno di legge, senza generare attese e illusioni negli abitanti dei territori interessati, senza, tra l'altro, incursioni del Governo fuori dalla logica istituzionale, come dimostrano le prese di posizione sulla stampa di oggi di autorevoli rappresentanti locali. Le Le risposte attese dalle popolazioni interessate, che peraltro hanno seguito il prescritto *iter* di legge, riguardano in estrema sintesi la relazione esistente tra territori cosiddetti ordinari e territori a Statuto speciale, con tutto il carico di disparità di trattamento economico e sociale, assurdamente e anacronisticamente garantito in Costituzione, che questo porta con sé. Proprio per cercare di affrontare e limitare le forti sperequazioni esistenti, soprattutto nei territori e nei Comuni confinanti con i territori speciali - in questo caso 28 Comuni del Veneto confinanti con il Friuli-Venezia Giulia - propongo di avviare la trattazione, il prossimo mercoledì, del disegno di legge n. 2279, concernente azioni e progetti a favore dei territori dei Comuni della Regione Veneto confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia,

Veneto. Il calendario procede con estrema regolarità. Abbiamo anche potenziato gli orari - ora andremo avanti fino alle ore 14 e la settimana prossima addirittura non avremo nemmeno gli orari di chiusura per le prime due giornate non si capisce perché estrapolare l'unico testo frutto di una indicazione territoriale successiva adei *referendum* popolari che chiedono di modificare dei confini.

di un *iter* che è già partito, che ha già visto le consultazioni popolari e le delibere delle Regioni (di distacco e di annessione).

Il collega Pegorer ha fatto capire che probabilmente, anche all'interno della maggioranza, non c'è la convinzione di procrastinare *sine die,* e speriamo che all'interno del PD tante persone rispettino almeno le volontà dei territori ai quali appartengono.

in poche ore. Abbiamo le ore di oggi. Abbiamo le ore di questa sera: che si incardini questa sera sul tardi o si incardini il terzo settore martedì mattina, non avremmo neanche gli emendamenti pronti perché li dovremmo presentare entro le

Il Parlamento non è stato minimamente informato. La Regione Liguria non è stata minimamente informata e men che meno lo sono state le attività economiche, e cioè i pescatori del posto, i quali si sono visti calare

Signor Presidente, com'è stato chiarito dal nostro vice Capogruppo, la Lega Nord voterà a favore di qualsiasi proposta che preveda il mantenimento in calendario

che vi siano provvedimenti più urgenti che meritano un'attenzione particolare o se, invece, la scelta della maggioranza e del capogruppo Zanda, a nome del Partito Democratico, è politica e allora avanzo la seguente proposta.

dei cittadini di Sappada, poi con un voto del Consiglio comunale, con un *referendum* plebiscitario, con un voto del Consiglio regionale del Veneto, con un voto del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con il voto delle Commissioni competenti del Senato della Repubblica. È inaccettabile che, di fronte alla manifesta volontà popolare degli organi istituzionali del nostro Paese, la Conferenza dei Capigruppo, per volontà della maggioranza, escluda l'esercizio di un diritto fondamentale, un diritto democratico che è quello delle comunità,

e aspettative in una popolazione che ha seguito le regole del vostro gioco, le regole del gioco dello Stato italiano, e che oggi si vede tradita in modo vergognoso dal comportamento della maggioranza. Se voi non credete politicamente alla bontà del provvedimento, non avreste dovuto inserirlo

La vera risposta alle istanze autonomiste sarebbe l'autonomia della Regione Veneto, ma almeno si conceda a chi ha seguito la regole del gioco di poter vedere rispettata la propria volontà. Chiedo veramente ad ogni singolo senatore di rivedere la decisione assunta nella Conferenza dei Capigruppo e di votare liberamente affinché il provvedimento venga democraticamente e responsabilmente votato in quest'Aula. *(Applausi

né è successo nulla di particolare. È stata una scelta democratica e legittima di quei Comuni. Oggi c'è un piccolo Comune che ha svolto tutte le procedure democratiche per arrivare a una risposta e sinceramente non si capisce perché il Senato non debba votare e ratificare la scelta di chi, credendo nelle istituzioni, ha fatto tutto quello che doveva fare per determinare la

Presidente, da uomo di confine, anzi, dei confini, credo sia giusto richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla delicatezza di interventi in questa materia. Ritengo che mettere mano ai confini delle Regioni e, in particolare, ai confini di quella Regione, che sono stati, per molti aspetti, tormentati e frutto di una storia in alcuni casi e per lungo tempo persino violenta, richieda una discussione e un approfondimento del tutto particolari. Sulla base di questa premessa, dico che condivido senza riserve la decisione della Conferenza dei Capigruppo, che propone una pausa di riflessione sull'argomento in questione. Si tratta di una posizione, la mia, che è frutto di un'antica esperienza politica e istituzionale. Mi considero un vecchio regionalista regionalista e anche un cultore della virtù della specialità dell'istituto regionale, che per lungo tempo ho contribuito a governare, stando sui banchi del Consiglio e anche intorno al tavolo della Giunta. Per tutte queste ragioni, mi pare che si debba apprezzare la decisione della Conferenza dei Capigruppo e anche la posizione che mi pare aver inteso sia del Governo, che propone sulla materia un'adeguata riflessione politica ed istituzionale.

provvedimento sul distacco di Sappada, un testo presentato dalla nostra ex collega Isabella De Monte, il cui *iter* è iniziato in Commissione il 22 ottobre 2013. Chi ha partecipato ai lavori della Commissione conosce

dopodiché a richiesta saranno restituite.

colleghi, non è possibile una pace onorevole con il nemico in armi all'interno dei propri confini. È questa la situazione del nostro Paese, dove le mafie ancora oggi martoriano tanti cittadini, a Nord e a Sud, gestendo o proteggendo militarmente attività illecite e dannose come la creazione e il rogo delle discariche abusive in Campania (penso alla terra dei fuochi) o sostituendosi allo Stato come garanti dei rapporti sociali ed economici nei quartieri degradati, fino a imporre comportamenti o a taglieggiare imprenditori. Ho sentito cittadini che hanno sporto denuncia contro reati comuni o finanziari o legati all'attività commerciale. A costoro è stato chiesto di ritirare le proprie denunce all'autorità giudiziaria e, di fronte al rifiuto, hanno iniziato un vero e proprio calvario. Lo Stato ha ancora molto da mettere in campo per accompagnare e sostenere chi denuncia. Chi ha denunciato spesso si sente solo di fronte alle organizzazioni criminali. Vedete, colleghi, la stragrande maggioranza delle nostre forze di polizia e della magistratura fa il proprio dovere ogni giorno, ma lo fa con fondi e mezzi scarsi, e le loro difficoltà si avvertono.

al più presto. Come al più presto devono essere portati in Aula i progetti di legge, come il disegno di legge n. 455, già presentato, per impedire di fare propaganda politica a persone sottoposte a sorveglianza per associazione mafiosa, disegno di legge che aspetta in Commissione dall'aprile 2016. Come al più presto deve essere rivisto il sistema di gestione dei beni confiscati alla mafia, a cominciare dalle liquidità e dal loro impiego, che devono essere messi, con urgenza e trasparenza, a disposizione della collettività per dimostrare che sono più fruttuosi se gestiti nella legalità. Ma, oltre all'operatività concreta, è fondamentale l'isolamento culturale delle mafie,

la consacrazione di valori positivi, a fronte dell'individualismo sfrenato e della sopraffazione che sottendono la cultura mafiosa. Chi ha avuto modo di stare in mezzo alla gente in un quartiere povero di qualche grande Città - come Palermo, Roma, Napoli e Milano - sa che lì spesso lo Stato è percepito solo come vessazione. La scuola e il supporto sociale, attento e rispettoso, sono fondamentali in luoghi come questi. Sono i primi avamposti dello Stato, quanto e più delle stazioni dell'Arma dei carabinieri e dei commissariati di polizia, com'è fondamentale l'opera di tante associazioni impegnate in questi contesti difficilissimi. Libera coordina tante di queste realtà e da venti anni celebra la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, realizzando attività volte a mantenere vivo il ricordo e la consapevolezza della velenosa concretezza delle mafie. Questo disegno di legge, che propone di istituire la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, può costruire una sutura importante tra l'impegno della società civile e l'impegno istituzionale su questo tema. Nel giorno del 21 marzo, data di inizio della primavera e per ciò stesso simbolo, nell'immaginario collettivo, di rinascita e di speranza, l'istituzione della giornata rappresenta un'occasione per restituire centralità nel dibattito pubblico al tema della lotta alle mafie, per promuovere la cultura della giustizia e della legalità, per responsabilizzare i giovani e stimolarli a un impegno personale nella difesa dei valori della convivenza civile. In questa giornata potranno essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, iniziative volte a costruire una memoria delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e le migliori pratiche poste in essere dallo Stato nella politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie. Dobbiamo acquisire una consapevolezza:

esso deve farsi carico anche di tutte quelle azioni concrete che descrivevo prima, dalla gestione dei beni confiscati, fatta in modo trasparente fino all'estremo, fino al parossismo.

ed è quella sorta di guerra civile sotterranea che di tanto in tanto affiora e si vive in tanti posti del nostro Paese.

e alto senso di responsabilità siamo qui riuniti oggi, con l'obiettivo comune di istituire una Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. È stato proposto, per questa importante occasione, il giorno 21 marzo, anche per dar seguito alla ventennale celebrazione organizzata da Libera, che scelse, nel lontano 1996, il primo giorno di primavera, quando il risveglio della natura diventa metafora di rinnovo di una primavera di verità e giustizia sociale, che dà fine ad un inverno di sofferenza e lutti. L'elenco, composto da oltre novecento nomi di vittime innocenti, che ogni anno, in una città diversa, viene letto in una solenne e commovente cerimonia, è servito per tenere vivo il ricordo, nei nostri cuori come in quelli di tante vedove, vedovi, genitori, figli senza padri, madri e fratelli, di vittime più conosciute, i nomi delle quali richiamano un'emozione forte, e meno conosciute, per le quali sentiamo il dovere civile e morale di ricordarli e tramandarli a futura memoria, offrendo inoltre sostegno morale ai loro familiari, in un momento condiviso di intensa riflessione. Voglio quindi rivolgere anzitutto un pensiero a tutti i familiari che con affetto e trasporto hanno contribuito a raccontare, in tutti questi anni, le storie di impegno civico e sacrificio proprie e dei loro cari. Dobbiamo far sì che questi straordinari esempi entrino definitivamente a far parte della nostra memoria collettiva. Un saluto inoltre anche alle tante associazioni, alle quali esprimo profonda gratitudine e riconoscenza, per l'incessante opera di difesa della memoria delle vittime. L'Italia - in particolare il suo Mezzogiorno - ha offerto un tributo di sangue e sacrificio continuo, dai primi del Novecento sino ad oggi. Ci sono le tante vittime cadute nell'esercizio del proprio lavoro o mentre erano alla ricerca della verità: membri delle Forze dell'ordine e della magistratura, che a testa alta, sprezzanti della paura e del pericolo, non si sono arresi alle minacce e alle intimidazioni, ma hanno rappresentato un baluardo dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, un fulgido esempio di virtù morale e passione civile. Ci sono poi tanti nomi di giornalisti, politici e membri della società civile che, non volendo piegarsi a regole non scritte di sottomissione e paura, hanno pagato con la vita l'aver tenuto la schiena dritta e l'aver raccontato, denunciato e combattuto un sistema che sembrava invincibile. Come non ricordare poi, tra le vittime di mafia, tutti i morti di tumore e altre patologie associate allo sversamento di rifiuti pericolosi e ai roghi di materiale tossico avvenute in Campania, in quella zona ormai tristemente nota come terra dei fuochi? pubblicati dall'Istituto superiore di sanità mettono in luce l'alto tasso di incidenza di tumori tra i bambini e gli adolescenti: a loro va la nostra solidarietà, ma anche la promessa che una cosa del genere non possa accadere mai più nel nostro Paese. Infine, voglio ricordare - anche loro non vanno dimenticati - i tanti cittadini caduti perché colpevoli solamente di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, durante un regolamento di conti o al momento dell'esplosione di un ordigno intimidatorio. Anche a loro dobbiamo mandare un ricordo affettuoso perché nel nostro Paese non si muoia più colpiti a sangue freddo perché lo Stato non riesce ad impedire faide e sparatorie alla luce del giorno e nei luoghi pubblici. pubblici. Signora Presidente, onorevoli colleghi, da cittadina, da senatrice e da membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, voglio ribadire che solo attraverso un'incessante operazione di recupero della memoria, di rafforzamento culturale e civile e di sostegno alle leggi e alla Costituzione del nostro Paese,

alla giustizia e introdurre misure di buona amministrazione per prevenire la delinquenza, combattendo il problema a livello territoriale e sociale. Poiché la peggior sconfitta per lo Stato avviene quando chi denuncia, chi non si volta dall'altra parte, chi urla ad alta voce che la mafia deve sparire, si sente solo ed abbandonato, questa Giornata deve essere un monito per ricordare a tutti che lo Stato c'è e fa il suo dovere prima di tutto e tutti. L'omertà, che troppo spesso è un ostacolo in questa lotta, diventa automaticamente un'alleata della mafia ed è contro di questa che dobbiamo batterci tutti, un Paese che è ancora imbevuto di cultura mafiosa, quella che molti commentatori definiscono sottocultura. Peccato, però, che chiamarla sottocultura non ci semplifica il compito, ma - anzi - lo rende ancor più angosciante. Come soleva dire Peppino Impastato, un'altra vittima eccellente che voglio ricordare (lasciata sola dietro i microfoni della sua Radio Aut, quando denunciava gli intrecci mafiosi della sua terra): «La mafia uccide, il silenzio pure». Poiché non vogliamo essere uccisi individualmente, né come comunità, nel nome e nella memoria delle tante vittime, sosteniamoci a vicenda in questa battaglia e teniamo la schiena dritta, come dritta è stata la schiena delle tante vittime che vogliamo ricordare. Se ogni cittadino manterrà vivo il ricordo, la mafia non avrà futuro.

Devo dire che il Parlamento esagera, secondo me, in una specie di santificazione laica dei giorni della memoria; ormai passiamo dal dal giorno del ricordo al giorno della memoria, alla giornata di quello e alla giornata di quell'altro. Non posso dimenticare, nel mio passato giovanile, quando la stessa cosa si cominciò a fare con la Resistenza:

dal generale De Lorenzo alla strage di piazza Fontana, fino al tentativo di golpe di Junio Valerio Borghese. Dico questo per dire che non dobbiamo correre il rischio di fare la stessa cosa con la mafia. Cerchiamo di essere chiari: oggi l'antimafia è in crisi. Oggi, se andate in giro o guardate attentamente i giornali, scoprirete che le polemiche sull'antimafia sono persino sono persino più forti del contrasto alla mafia. Il sospetto investe alcuni personaggi; ci sono imprenditori che sollecitano il distintivo antimafia e che però sono in odore di mafia (è successo in Sicilia). Lo stesso scioglimento - ne abbiamo parlato ieri in Commissione - di alcuni Comuni diventa oggetto di battaglia politica e l'accusa «tu non hai le carte in regola» anch'essa diventa oggetto di battaglia politica. In certi momenti anch'io, che lo criticai all'epoca, sento riecheggiare nella mia testa le parole di Leonardo Sciascia sui professionisti dell'antimafia.

è difficile che un dirigente antimafia non abbia un forte carattere e che poi, certo, è quasi impossibile metterne due o tre insieme. Quindi siamo semmai in un periodo in cui la celebrazione non giova, mettiamola così. E non giova neanche far finta di avere tutte le carte in regola. Ho sentito il procuratore antimafia, in una recente occasione, dire che a questo punto corriamo il rischio di contenere

se abbia ancora senso una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso. Sapete, colleghi, le Commissioni parlamentari di inchiesta dovrebbero durare fino a chiarire qual è il fenomeno e a proporre delle iniziative straordinarie per contrastarlo. Se diventano permanenti, le Commissioni parlamentari bicamerali

Un sindaco - non dirò quale, per evitare lo scontro di un partito contro un movimento, che potete immaginare - è stato chiaramente oggetto di un'intimidazione mafiosa con ricatto, perché è venuto un suo consigliere e gli ha detto: «Qui c'è la prova di un abuso. Mettila in cassaforte e assumi questo». Questo sindaco ci ha detto: «Ma, sai, non c'erano le minacce esplicite e quindi non c'era la fattispecie del reato». Capite che noi continuiamo a parlare di mafia, anche all'interno della Commissione antimafia, cancellando tutta l'esperienza dello studio e del contrasto alla mafia. È evidente, infatti, che la minaccia si fa proprio così. Diceva sempre Pif, in questo pezzo che pubblico sulla rivista «Left»: rivista «Left»: «Noi eravamo seduti per strada a Palermo, il tavolo molto vicino alle macchine. Ad un certo punto uno, un po' più arrogante, si è messo a suonare il clacson. Il mio amico di Reggio Emilia ha detto: "È quello il mafioso". E noi palermitani gli abbiamo detto: "No, no, non è quello il mafioso. Il mafioso sarebbe stato gentilissimo, mai arrogante, avrebbe chiesto scusa"». Ecco, vedete, è evidente. Chi conosce la mafia sa che la mafia è un potere intollerabile ed assurdo, ma non è da confondersi con il bullo. E il fatto che non ci sia la fattispecie del reato non vuol dire assolutamente niente, perché l'intimidazione di mafia si sa e si deve riconoscere. Questo lo dico perché le celebrazioni mi lasciano molto perplesso. Se fossi in questo Parlamento, invece di riempirmi la bocca con l'antimafia starei a sentire le parole sante del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, ogni volta che parla, inascoltato, pone la questione su un altro fenomeno, che è generatore della mafia,

quanto stiamo facendo tuttora. Invece, è troppo facile prendersela con i *killer*, che carichiamo di ergastoli, che teniamo in quelle condizioni, senza poi vedere, invece, chi sfrutta una certa retorica dell'antimafia per continuare a fare i suoi affari. Ci sono stati casi che non cito. C'è stato anche un sindaco antimafia che dava i soldi ai parenti dei mafiosi perché parlassero con i loro congiunti in carcere, anche superando le normative di restrizione e altri esempi di questo genere. di questo genere. Faccio questo intervento perché ritengo che in Parlamento bisogna dire la verità. Non ci si schiera soltanto; bisogna dire la verità

di far camminare l'antimafia sulle gambe di tanti ragazzi e delle famiglie che sono state spesso dimenticate dallo Stato, non ascoltate e non valorizzate quando erano disposte a evocare il sacrificio dei loro congiunti per fare qualcosa. Parlo di tutte le famiglie e non soltanto di quelle delle vittime illustri della mafia; di tutte le vittime della mafia. Ogni anno il 21 marzo, il primo giorno di primavera, c'è questa manifestazione che Luigi Ciotti organizza. È stata bellissima nel 2015; ora sarà un po' diversa e quest'anno sarà a Messina.

anche noi questa Giornata è un modo - nella mia testa almeno - di uscire dal palazzo, di aprire le porte e far entrare un po' di aria e, quindi, voterò a favore di questa istituzione. Signora Presidente e onorevoli colleghi, oggi discutiamo un disegno di legge breve e forse anche solo simbolico: e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. È una legge importante, pur se simbolica. Con la mafia siciliana, la 'ndrangheta calabrese, la camorra campana e le altre mafie italiane i simboli sono importanti. Servono a ricordare e a ribadire dove sta il bene e dove sta il male. Sono manichea? Ebbene sì. Con le mafie non c'è scelta: si combattono o si sceglie la complicità. Potrei parafrasare Tolstoj, nell'inizio di Anna Karenina; mentre la lotta alla mafia si fa in modi che si somigliano tutti, dicendolo e facendolo tutti i giorni, inflessibilmente, la contiguità e la complicità hanno molte manifestazioni diverse, quali l'omertà, l'oblio, la sciatteria amministrativa e intellettuale, l'opportunismo. Leggi come queste servono a distinguere chi si è battuto con coraggio e schiettezza contro la criminalità ed è stato ucciso dalle mafie da chi invece è rimasto a guardare, per indifferenza, codardia o per convenienza. Isaia Sales, nel suo recente e bel libro «Storia dell'Italia mafiosa» ricorda come Giulio Andreotti non andò al funerale di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quando gliene chiesero conto lui rispose: «Preferisco i battesimi ai funerali». di farci da guida e da faro nei tempi bui del grigiore burocratico che offusca la memoria del male mafioso e del bene di chi lo combatte.

Perché - Presidente e Governo - quella proposta è ferma in Commissione giustizia? Perché non fa passi in avanti la riforma, pur compromissoria, della prescrizione? Perché consentiamo agli avvocati dei mafiosi di tirare a guadagnare l'estinzione del reato per prescrizione fino in Cassazione, in modo da assicurare loro l'impunità? Vedete, Presidente e colleghi, il 22 dicembre 2015 la Corte di cassazione ha depositato la sentenza su Rosario Perri, il direttore dell'ufficio tecnico del mio Comune, che aveva rapporti con la locale di 'ndrangheta di Desio e con il suo vertice, Annunziato Moscato, condannato a sua volta nell'ambito dell'indagine denominata Infinito. Il reato di Perri è stato dichiarato prescritto, pur avendo la Cassazione scritto parole inequivoche e definitive che egli abbia commesso quel fatto-reato. Ora, il Comune di Desio ha deciso di proporre azione civile per il danno da reato per ben 7 milioni di euro. Penso che in un Paese civile un reato grave contro la pubblica amministrazione non possa prescriversi così facilmente, tanto più se questi reati sono il brodo di coltura degli interessi delle mafie.

Oggi e ogni giorno, nel nostro Paese, c'è una storia da ricordare: una storia intrisa di dolore, che racconta di vite spazzate via dalla mano vile di chi utilizza la violenza per ottenere vantaggi personali in modo prepotente e illegale. storie di uomini e donne che hanno scelto di stare dalla parte della legalità, pagando magari un prezzo altissimo. Per i familiari che hanno vissuto tali situazioni ogni giorno è un riaffiorare di dettagli e di ricordi che uccidono ancora: nomi, fotografie, articoli sui giornali, processi nelle aule dei tribunali. Storie di una quotidianità, di famiglie, di affetti annullati per sempre. È un dovere morale, per chi resta, mantenere viva la memoria di chi non c'è più, ma lo è ancora di più per le vittime innocenti di mafia. Diventa una sorta di "urgenza'", signor Presidente, per i familiari delle vittime mantenere viva almeno la memoria di chi è stato ucciso in nome della dignità, dell'onestà e per affermare la legalità. Come esponenti della Lega Nord non possiamo non ricordare, tra le vittime della mafia, anche le vittime della tratta di esseri umani, compiuta da trafficanti senza scrupoli, che hanno trovato appoggi e collusioni con esponenti della criminalità organizzata nel nostro Paese.

ricordare al Governo che anche in questo caso contro la mafia si sta facendo poco. In questa giornata tutte le vittime di mafia saranno uguali e urleranno la stessa sete di giustizia; servirà a far vergognare esecutori materiali e mandanti, servirà a trasmettere un po' di forza e di coraggio ai tanti magistrati che ogni giorno subiscono tutte le difficoltà della lotta Ricordo sempre che qualche volta qualcuno si aspetta ancora il mafioso come l'uomo che indossa la coppola e la lupara, ma non è più così. Ricordare è importante, ma lo è ancora di più conoscere la verità sulle stragi che hanno insanguinato questo Paese e che restano ancora senza risposta e senza responsabili. sono state circa 1.120 le vittime innocenti di mafia che lacerano, come un profondo taglio, oltre cento anni di storia di questo Paese. donne, ragazzi, bambini, pensionati che per sbaglio o per precisa volontà delle cosche finiscono trucidati per questioni ben più grandi di loro. Chissà quanti di cui non si ha memoria saranno finiti nell'oblio di un archivio polveroso in un remoto paese di provincia o saranno covati o tenuti nascosti dai famigliari come un dolore troppo grande da rendere pubblico. Si deve rendere onore alla memoria dei caduti in servizio di tutte le Forze dell'ordine, cioè di coloro che hanno sacrificato la loro vita, rimanendo vittime di atti terroristici o di azioni criminali per mantenere alto lo spirito democratico di libertà. Sono da considerare vittime del dovere gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia penitenziaria, alle Polizie municipali e al Corpo nazionale del vigili del fuoco. È necessario rendere giustizia a tutti quei morti e ai loro famigliari. chi ha sbagliato deve pagare e lo deve fare con pene certe, senza condoni. Solo così potremo davvero onorare chi ha sacrificato, spesso consapevolmente, la propria vita per un futuro migliore e per affermare con coraggio la legalità. Lo Stato deve essere in grado di compiere azioni per riconoscere e ricordare in modo degno quanti hanno sacrificato la loro vita per la società civile e per la nostra sicurezza. Il calo degli omicidi di mafia e di conseguenza del numero di vittime innocenti registrato a partire dagli anni Duemila è una buona notizia, ma questo dato

come testimoniano i 130 Consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose negli ultimi quindici anni. La mafia non esita a uccidere donne e bambini: la morte è l'unica legge che conta e di cui è padrona. Sono 124 le donne innocenti uccise da mani mafiose in Italia e 105 sono stati i minorenni, tra cui bambini e a volte bimbi piccoli di pochi Per molti anni si è venduto il cosiddetto codice d'onore mafioso come qualcosa di parallelo e di positivo, ma forse questa positività era più degna delle pellicole cinematografiche; poi si analizzano i dati, si piange e si arriva alla conclusione che la criminalità mafiosa non risparmia nessuno. Pensiamo a tutti quei casi in cui donne e bambini si sono trovati a essere vittime casuali, ma in cui in realtà la casualità

il 21 marzo, istituzionalizzando così l'iniziativa di Libera, che già da anni ha adottato il primo giorno di primavera come simbolo della battaglia sociale per mantenere vivo il ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata. o dovremmo sapere che non è consentito a nessuno di restare neutrale quando da una parte c'è chi infligge la violenza e, dall'altra, chi la subisce;

che abbiamo dimenticato. «Vittima» indicava l'essere vivente puro e innocente, sacrificato agli dei, ed esprimeva la storia di chi subisce la violenza senza colpa, in modo imprevisto e imprevedibile, soprattutto senza possibilità di sottrarsi. È vittima non solo chi subisce la violenza sulla sua carne, ma anche chi gli sta accanto e patisce la perdita e la conseguenza dell'ingiustizia. I nostri esperti antimafia si sono convinti negli anni che la migliore lezione di legalità - e quindi di antimafia - sia far funzionare la Repubblica. Tanto meglio funziona la Repubblica, tanto meno c'è bisogno di mafia. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa disse che la battaglia che dobbiamo combattere è complessa. «Lo Stato batterà la mafia quando assicurerà come diritti ciò che i mafiosi elargiscono come favori». Dall'altra sponda, da quella mafiosa, le parole del *boss* Pietro Aglieri, che disse a un magistrato: «Vede, dottore, quando voi andate nelle scuole e parlate ai nostri ragazzi, quelli, sì, vi ascoltano. Ma quando poi escono e cercano un lavoro, da chi vanno? Vengono da noi». Questa storia racconta e dice che la memoria è importante e l'impegno nel ricordo lo è altrettanto: vanno entrambi tenuti vivi. Cosa sapremmo dell'Olocausto se a raccontarlo fosse stato qualche boia tedesco e non il deportato 174 517. È così anche per le vittime innocenti della mafia e del terrorismo e di ogni grave ingiustizia. *(Applausi dei

Non basta più affidare ai singoli, tra l'altro spesso lasciati soli, la lotta alle mafie. Le mafie si possono sconfiggere: va detto soprattutto in queste Aule; va detto da tutte le istituzioni e in ogni intervento. Va usato il potere che abbiamo di legiferare per dire che le mafie si possono sconfiggere. non viene più presa in considerazione: sembra che le mafie esistano, si debbano lasciare esistere e, anzi, si debba scendere a compromessi con loro. Invece è ora di dire basta ai compromessi e ai giochi al ribasso. Le mafie si possono sconfiggere e deve diventare un *mantra*. Noi abbiamo qui il dovere e il potere di dimostrare che le mafie si possono sconfiggere. Non basta più la commemorazione e la memoria: dobbiamo fare qualcosa per evitare di dover poi commemorare le vittime di mafia, alle quali ovviamente va il nostro ricordo e il sostegno alle famiglie. Ma in queste Aule dobbiamo tenere presente che le mafie si possono e si devono sconfiggere. Noi le possiamo sconfiggere e quindi dobbiamo fare in modo, con il potere di legiferare che abbiamo, di sconfiggerle ogni giorno, in tutte le nostre azioni compiute in queste Aule. Basta con le commemorazioni: atti concreti. Sconfiggiamo le mafie.

poco conosciuta, ma non per questo meno importante. La suddetta Commissione, posta a tutela, in chiave preventiva, dei beni ambientali fu voluta dall'Unione europea dopo l'approvazione di un analogo atto, verso la fine del 1969, dal Congresso Nello specifico, la valutazione di impatto ambientale nazionale viene introdotta in Italia sulla base di norme transitorie che traggono origine da quanto definito dall'articolo 6 della legge n. 394 del 1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente e conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 1985, modificata ed integrata dalla direttiva CEE n. 97 del 2011. Secondo la normativa comunitaria, i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso come ambiente naturale e e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Questa può essere nazionale o regionale in base a determinate categorie progettuali. Essa si struttura su più livelli: la VIA vera e propria, la VAS (valutazione ambientale strategica), l'AIA (autorizzazione ambientale integrata), la VIA speciale (valutazione opere della cosiddetta legge obiettivo, le grandi opere della legge Lunardi n. 443 del 2001). La sua funzione, pertanto, è assolutamente strategica, soprattutto per quei territori, come l'Italia, soggetti ad uno strutturale ed endemico pericolo di dissesto idrogeologico

nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti ed esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche con adeguata qualificazione in materie tecnico-ambientali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 luglio 2007, poi, sono stati stabiliti il funzionamento e l'organizzazione della commissione medesima. Nella sostanza, la commissione VIA è l'organo pubblico che decide se un'opera si può fare o no. Vi è, però, un problema. È noto come, infatti, molti dei suoi componenti lavorino per aziende private i cui affari dipendono direttamente dai pareri dei commissari: un'anomalia che il Governo non ha risolto, nonostante più volte sollecitato Pertanto, risulta alquanto difficile, se non impossibile, parlare d'imparzialità. Non sembra, infatti, plausibile che i commissari VIA, chiamati ad esprimere i pareri su grandi opere pubbliche, quali - a titolo meramente esemplificativo - la TAV, possano nutrire interessi privati.

così come del resto il presidente del Consiglio Renzi. Pertanto, ritengo utile accendere i riflettori sulla commissione in questione, sottolineando la necessità di procedere al rinnovo della medesima, in quanto la stessa, più volte prorogata e scaduta ormai dal giugno 2014, si ritrova ad oggi in *standby*, e al contempo